Signora Presidente, la Farnesina, l'ambasciata d'Italia a Tokyo e il consolato generale d'Italia a Osaka conoscono bene e seguono con grande attenzione la vicenda segnalata dall'onorevole interrogante, fornendo assistenza al connazionale e ai piccoli nati dal matrimonio con una cittadina giapponese. Da quanto risulta alla Farnesina, il nucleo familiare, dopo aver vissuto per alcuni anni in Germania, si è trasferito - di comune accordo - in Giappone, a Tokyo, nell'ottobre 2015. Pochi mesi dopo, tuttavia, a causa del deterioramento del rapporto coniugale, la madre dei piccoli è tornata a Nagasaki, sua città natale, portando con sé i bambini. allora la cittadina giapponese ha reso molto difficile il rapporto tra il padre e i figli, ostacolandone i contatti. È attualmente in corso in Giappone un procedimento giudiziario per definire i termini della questione, nell'ambito del quale il connazionale ha conferito mandato a un legale che lo difenda e lo assista. Al riguardo, la sentenza sarà pronunciata probabilmente entro la prima metà del prossimo mese di novembre. Il 28 aprile scorso si è tenuta la terza udienza presso il tribunale dei minori di Nagasaki che ha portato alla concessione al padre del diritto di visita ai minori. Si tratta di un'evoluzione positiva del contenzioso familiare; il 2 giugno scorso il connazionale ha quindi potuto incontrare i suoi figli e il 29

grazie L'ambasciata d'Italia a Tokyo e il consolato generale a Osaka, d'intesa con la Farnesina, hanno più volte tentato una mediazione tra i coniugi, alla ricerca di una soluzione che contemperi le reciproche pretese genitoriali con il diritto dei minori a preservare il rapporto con entrambi i genitori. Il connazionale è stato più volte accolto in ambasciata, da ultimo lo scorso 5 ottobre, dove ha trovato sempre ascolto e partecipe attenzione. Di recente, poi, nell'ambito delle periodiche riunioni di coordinamento consolare in ambito europeo, l'ambasciata ha poi avviato un giro d'orizzonte con gli altri *partner* europei accreditati a Tokyo per valutare e discutere casi simili a quello che coinvolge il nostro connazionale, con l'obiettivo di condividere le esperienze di tutela consolare e scambiare informazioni utili.

Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Faraone, che mi ha permesso di avere la risposta in Assemblea alla mia interrogazione. Devo dire, quindi, non tanto al Sottosegretario, quanto alla Farnesina che fornisce questi dati, che la risposta se, da un lato, mi rinfranca rispetto al fatto che il Ministero degli affari esteri si sia attivato

Signora Presidente, prima di passare al merito dell'atto ispettivo in esame, desidero ricordare che lo stesso, presentato pochi giorni prima dell'incontro dei Capi di Stato e di Governo del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7) che ha avuto luogo a Taormina il 26 e 27 maggio scorsi, era stato posto da subito nella programmazione del sindacato ispettivo di quest'Assemblea, in modo tale da fornire un'informazione tempestiva al senatore interrogante. Rispondere oggi, a evento terminato, risulta comunque particolarmente opportuno - e per questo ringrazio il senatore interrogante - poiché rende possibile illustrare in quest'Assemblea l'insieme delle misure di organizzazione sanitaria di specifica competenza regionale che hanno concorso all'ottima riuscita organizzativa dell'evento, contribuendo, anche per questo verso, alla diffusione di una positiva immagine internazionale del nostro Paese. Come noto, la portata dell'evento ha richiesto, accanto alle imponenti misure di sicurezza, una pianificazione specificamente rivolta

appartenente a diversi enti e istituzioni, che hanno contribuito, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a garantire il sereno svolgimento dell'evento. Per la realizzazione della pianificazione e delle conseguenti procedure operative, l'assessorato ha compiuto un lavoro di programmazione a carattere regionale, con l'obiettivo di fronteggiare al meglio le eventuali situazioni di rischio, anche nei loro aspetti evolutivi. In tale contesto, sono stati potenziati il sistema del soccorso territoriale del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica (118), con postazioni fisse e mobili diffuse in tutto il territorio regionale e a livello locale, per poter garantire la rapidità di intervento in qualunque area; il presidio ospedaliero di Taormina, di pertinenza all'azienda ospedaliera provinciale di Messina; i presidi ospedalieri di Messina e Catania, considerata l'equidistanza della zona di intervento rispetto ai due capoluoghi, nonché il servizio di eliambulanza nelle ventiquattro ore, dedicata all'evento G7. Inoltre, in considerazione della dimensione del vertice internazionale, il piano di assistenza socio-sanitaria si è prefisso di garantire, in particolare, l'assistenza sanitaria sia di base, che in emergenza-urgenza, ai Capi di Stato e di Governo alle loro delegazioni; il pronto arrivo dei soccorsi sanitari, con percorsi dedicati, a vantaggio della popolazione residente nella zona interessata dall'evento; l'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza e i relativi trattamenti in caso di manifestazioni e di eventuali attentati; infine, l'assistenza sanitaria a tutto il personale temporaneamente operante nel territorio. La pianificazione curata dalla Regione Siciliana, oltre alle risorse umane, ha coinvolto diverse strutture ospedaliere ubicate nel territorio provinciale di Messina e Catania, poste nel massimo stato di attenzione e pronte all'attivazione del prestabilito piano di emergenza interno per massiccio afflusso di feriti. Tale rete di assistenza sanitaria ha previsto un sistema di soccorso in grado di consentire, in caso di necessità, la massima rapidità d'intervento e la debita riservatezza a vantaggio dei partecipanti all'evento internazionale.

anti G7. Esso pertanto, dipendente dall'azienda sanitaria provinciale n. 5 di Messina, è stato potenziato fino alla massima capacità ricettiva e interventistica e, per il periodo d'allerta dell'evento, apprestato anche alla procedura delineata nel piano di emergenza interno per evacuazione. Nei riguardi della popolazione residente, la stessa pianificazione regionale ha previsto che, in ogni eventuale caso di richiesta d'attivazione dell'assistenza sanitaria al 118, l'ospedale di riferimento sarebbe stato il San Vincenzo di Taormina. Quest'ultimo infatti, anche nei giorni dell'incontro internazionale, ha continuato ad ospitare i pazienti già assistiti, mentre ha sospeso unicamente i ricoveri programmati, rimanendo, in ogni

che ha riguardato una donna extracomunitaria, la quale aveva da poco partorito una neonata a bordo della nave Libra della Marina militare italiana, diretta al porto di Reggio Calabria e che, in quel momento, navigava al largo della costiera di Giardini Naxos. La donna e la neonata facevano infatti parte di un gruppo di 472 migranti salvati nel Canale di Sicilia, e sono state portate a terra da una motovedetta della capitaneria di porto e quindi trasportate all'ospedale. Concludo pertanto rassicurando il senatore interrogante che lo svolgimento del G7, nel richiedere certamente un potenziamento della rete assistenziale siciliana collegato alle peculiari esigenze dell'evento, non ha comunque pregiudicato l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che sono stati garantiti alla cittadinanza senza determinare sospensioni o interruzioni tali da compromettere la salute dei pazienti.

mi ha impedito di rassicurare quanti mi avevano segnalato i timori che ho rappresentato con l'interrogazione per tempo. Ad oggi, mi fa piacere avere una rappresentazione dell'operatività posta in essere in quei giorni, ma la preoccupazione, in assenza di risposte,

siamo messi maluccio, considerato che, su 146 interrogazioni che ho presentato in questa legislatura, ho ricevuto 39 risposte (inclusa questa). È quindi da immaginare che negli altri casi il Governo abbia ritenuto più opportuno per la propria immagine politica non rispondere.

la situazione della sanità in Sicilia francamente è assai carente, soprattutto per quanto riguarda le strutture di pronto soccorso.

bene. Devo dire, tuttavia, che è normale per chi abiti in Sicilia, anche nelle grandi città, ritrovarsi davanti a strutture di pronto soccorso gremite oltremodo, con tempi di attesa,

Questo aspetto è legato sicuramente a una carenza di fondi per la sanità che, da quello che ho avuto modo di leggere nel DEF, che è stato da poco approvato, approvato, vanno incontro a una continua decurtazione. La cosa avrebbe un senso politico più facilmente comprensibile se tale decurtazione si accompagnasse e conseguisse a una riduzione delle inefficienze. L'impressione, invece, che si ha è che le inefficienze siano quelle più dure a essere rimosse e che la riduzione dei fondi disponibili alla fine si sostanzi in una riduzione del servizio *tout court* che va a svantaggio degli utenti in un settore che, come lei può immaginare, è assolutamente cruciale nella vita di una persona.

presso la XII Commissione della Camera dei deputati, una dettagliata informativa in merito allo stato dell'emanazione del regolamento sull'erogazione del risarcimento dovuto alle vittime da talidomide. L'attività del Ministero, comunque, è proseguita incessantemente, anche in considerazione della rilevanza rivestita dalla tematica in esame che, come accennato, vede destinatari centinaia di persone affette dalla sindrome da talidomide. Pertanto, mi accingo a fornire gli ulteriori aggiornamenti relativi all'attività svolta dal Ministero proprio in questi ultimi giorni. Come ricordato dagli onorevoli interroganti, l'articolo 21*-ter* del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito dalla legge n. 160 del 2016, ha integrato la normativa vigente in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Tale disposizione, in estrema sintesi, ha esteso il diritto al riconoscimento degli indennizzi ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, anche ai nati negli anni 1958 e 1966, nonché ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo previsto dalla legge medesima, presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. In tale ultimo caso, tuttavia, al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, la legge ha previsto che, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporti le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 163 del 2 ottobre 2009, provvedendo in particolare a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti richiedenti. Fatta questa necessaria premessa - utile per comprendere fin da subito la complessità, innanzi tutto tecnico scientifica, del compito assegnato al Ministero della salute passo subito al merito del quesito posto per illustrare l'attività svolta finora da questa amministrazione. In considerazione della necessità di un esame approfondito e multidisciplinare degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide, ai fini della definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni per l'accertamento del diritto all'indennizzo a vantaggio dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, il Ministero della salute ha chiesto al Consiglio superiore di sanità - organo consultivo tecnico del Ministro della salute - di esprimersi in merito alla definizione dei predetti criteri e, in particolare, circa l'individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Il 17 gennaio 2017 le sezioni congiunte congiunte II e V del Consiglio superiore di sanità hanno espresso il parere sui criteri di inclusione ed esclusione, e, in particolare, sulla individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i nati fuori dal periodo 1958-1966. Tenendo conto della normativa intervenuta e del parere reso dal Consiglio, questo Ministero ha predisposto uno schema di regolamento. La bozza di regolamento è stata trasmessa al Consiglio superiore di sanità - deputato, tra l'altro, ad esprimere parere obbligatorio sui regolamenti che interessano la salute, ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1993 per la verifica della coerenza del predetto schema con l'avviso espresso dal Consiglio il 17 gennaio 2017 e per ottenere il parere. Le sezioni congiunte II e V del Consiglio superiore di sanità hanno reso in data 13 giugno 2017 il parere obbligatorio. A seguito delle osservazioni espresse nel parere del Consiglio superiore di sanità, il Ministero ha modificato in senso conforme la bozza di regolamento. In data 3 agosto 2017, il Ministero della salute ha richiesto il parere, ai sensi della legge n. 400 del 1988, al Consiglio di Stato, reso all'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017. Il parere favorevole con osservazioni e condizioni è stato spedito a questo Ministero in data 4 settembre 2017. Tra le condizioni di carattere generale poste dal Consiglio di Stato devo evidenziarne una in particolare: quella relativa alla tecnica normativa utilizzata per dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 21-*ter*. La scelta regolatoria di questo Ministero era stata, infatti, quella di riscrivere *in toto* il regolamento, apportando al medesimo le modifiche necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni legislative: ciò all'esclusivo fine di pervenire ad una migliore comprensione della regolamentazione a beneficio dei destinatari del provvedimento. Per quanto il Consiglio di Stato abbia molto apprezzato la scelta di questo Ministero di conferire maggiore chiarezza al testo, riscrivendo integralmente il regolamento con le modifiche necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni legislative, devo tuttavia rimarcare che l'alto consesso ha ritenuto necessario che l'intervento di aggiornamento dovesse avvenire interpolandone le disposizioni e, dunque, con il metodo della novellazione. Pertanto, è stato redatto il nuovo schema del regolamento che recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato e lo stesso è stato inviato lo scorso 28 settembre, secondo la raccomandazione del medesimo Consiglio di Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle necessarie verifiche in relazione agli oneri aggiuntivi che devono trovare copertura nei mezzi finanziari predisposti dalla legge. A seguito della verifica positiva effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, il 3 ottobre lo schema di regolamento è stato comunicato, così come prescritto dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, nel prendere atto della comunicazione, ha effettuato alcune osservazioni in data 9 ottobre 2017, le quali sono state accolte nella formulazione finale del regolamento. Posso, pertanto, rassicurare i senatori interroganti che l'*iter* previsto dalla normativa vigente per la redazione del regolamento si è concluso e che a breve potrà essere emanato e dunque pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

è che alla nuova riformulazione del regolamento corrisponda anche la possibilità di una dilatazione dei tempi di presentazione dell'indennizzo, strumento necessario per consentire alle persone che hanno il diritto di farne richiesta di avere più tempo rispetto alla data attualmente stabilita, che è quella del 28 dicembre. Presidente, esprimo soddisfazione per la definizione dell'*iter* e quindi per la prossima emanazione del regolamento.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, tengo preliminarmente a precisare che il Ministero presta la massima attenzione al tema delle imprese colpite da eventi atmosferici avversi. Per questo ringrazio gli onorevoli interroganti che hanno permesso di affrontare la tematica anche in quest'Aula. Proprio per questo e in considerazione dell'eccezionalità degli eventi richiamati dall'interrogante, abbiamo sostenuto e approvato l'emendamento alla manovra correttiva dei conti pubblici, che prevede una disposizione a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, nonché dalla siccità del periodo estivo, estendendo ad esse la possibilità di accedere ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale anche per le colture assicurabili. Con legge n. 123 del 2017 di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017 è stata approvata una modifica normativa voluta da questo Ministero che consente l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale anche alle imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici avversi in parola. La disposizione tiene conto del fatto che, sebbene gli eventi considerati siano assicurabili per la totalità delle colture vegetali, nelle aree maggiormente colpite dalle avversità segnalate gli strumenti assicurativi agevolati sono invece scarsamente utilizzati dagli agricoltori i quali - in caso di eventi eccezionali - non potrebbero contare su alcuna forma di compensazione, rischiando di vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva dell'attività. In questa prospettiva ricordo che il Fondo di solidarietà nazionale promuove interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole a fronte dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, per il ripristino dei danni alle strutture aziendali agricole, causati da calamità naturali o eventi eccezionali. Grazie a ciò, le aziende colpite dalle gelate o dalla siccità e che non abbiano sottoscritto polizze assicurative, potranno accedere ai benefici previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 per favorire la ripresa dell'attività produttiva. Le Regioni interessate potranno deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il 31 dicembre 2017, costituendo questo il presupposto per l'operatività delle misure. È stato predisposto ed è in corso di perfezionamento il decreto di declaratoria per le province di Vicenza e Verona per i danni alle produzioni causati in alcuni territori provinciali dalle gelate di aprile 2017. Questo Ministero, inoltre, per garantire maggiore liquidità alle imprese agricole, ha chiesto alla Commissione europea di autorizzare l'erogazione di anticipi almeno fino al 70 per cento per i pagamenti diretti e fino all'85 per cento per il sostegno concesso nell'ambito delle misure a superficie dello sviluppo rurale, nonché di applicare una deroga sul *greening* che consenta agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo e lo

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 2017 e sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - la cui misura 4 prevede espressamente «investimenti in infrastrutture irrigue», è scaduta lo scorso 31 agosto. Le domande sulle quali si è conclusa la fase istruttoria della verifica di ricevibilità contano un aiuto complessivo richiesto pari a euro 1.048.228.790,63. Le risorse a disposizione corrispondono a circa 600 milioni, con 300 milioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2015-2020 per realizzare grandi opere infrastrutturali irrigue e altri 295 milioni con il Fondo sviluppo e coesione. A questi investimenti si aggiungerà il finanziamento - da parte del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge recante il bilancio previsionale dello Stato, per l'anno finanziario 2017 per circa 106 milioni di euro, per sei progetti strategici, in quanto capaci di risolvere importanti criticità quali il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale, nonché la facilitazione di soluzioni di questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, va, preliminarmente, segnalato come la legislazione di settore e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, affidi la competenza primaria nella materia della lotta attiva contro gli incendi boschivi alle Regioni, riservando allo Stato il solo concorso nell'attività di spegnimento. La legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 ha, tra l'altro, attribuito alle Regioni il compito di definire e programmare, mediante appositi piani regionali, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In tale contesto, il Ministero dell'ambiente ha diretta competenza in materia di incendi solo con riferimento ai piani antincendio boschivi delle aree protette statali, mentre resta la diretta competenza delle Regioni nella lotta attiva, anche all'interno delle suddette aree protette. A tutela delle stesse, il 12 luglio scorso, il Ministero dell'ambiente ha emanato apposita direttiva nella quale sono incluse anche raccomandazioni

e/o aggiornare il relativo catasto. L'aggiornamento dovrà essere comunicato anche all'ente gestore per l'aggiornamento annuale del proprio piano Inoltre, nella consapevolezza che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenti una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese, il 5 aprile scorso è stato firmato un apposito protocollo d'intesa tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di definire ogni utile sinergia operativa e di migliorare ulteriormente l'efficacia degli interventi. Il 4 maggio 2017 è stato, peraltro, sottoscritto un apposito accordo quadro tra il Governo e le Regioni, il quale integra ulteriormente il quadro delle iniziative assunte per prevenire, per quanto possibile, su tutto il territorio nazionale, eventuali disfunzioni operative in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Il Ministero dell'interno ha evidenziato, altresì, che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale recante disposizioni attuative per l'istituzione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, ha adottato i provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo n. 177 del 2016. In particolare, ha provveduto ad inquadrare il personale del Corpo forestale effettivamente trasferito al medesimo Ministero dell'interno nei nuovi ruoli AIB ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A ciò si aggiunga che, a seguito del trasferimento del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato, sono stati istituiti i nuovi reparti di volo di Cecina, Lamezia Terme e Rieti. Inoltre, sin da gennaio, sono state attivate con l'ENAC le procedure per il mantenimento delle condizioni di aeronavigabilità dei mezzi aerei transitati dalla forestale al Corpo nazionale. La grave crisi ambientale verificatasi durante la stagione estiva, caratterizzata dalla diffusione di numerosi ed estesi incendi boschivi, oltre che da una prolungata siccità, ha determinato, peraltro, una protratta condizione di rischio per la conservazione della fauna selvatica in ampi settori del nostro territorio. Alla luce di tale situazione, l'esercizio dell'attività venatoria a carico di talune specie può rappresentare un ulteriore motivo di aggravamento delle condizioni demografiche delle popolazioni interessate, non solo nelle aree percorse dagli incendi, ma anche nei settori limitrofi e interclusi allorquando l'azione del fuoco abbia interessato percentuali importanti del territorio e quando gli incendi si siano succeduti nell'arco degli ultimi anni negli stessi comprensori. Si ritiene pertanto necessaria l'adozione di misure di limitazione del prelievo sulla base delle risultanze di specifiche iniziative di monitoraggio soprattutto a carico delle popolazioni di fauna selvatica stanziale o nidificante, potenzialmente oggetto di prelievo venatorio. In particolare, si ritiene utile un'estensione per almeno due anni del divieto di caccia in tutte le aree percorse dal fuoco, come già previsto dalla legge n. 353 del 2000 per le sole aree boscate, nonché ad una fascia contigua alle aree medesime, le cui dimensioni devono essere stabilite caso per caso in funzione delle superfici incendiate, della loro distribuzione e delle caratteristiche ambientali delle aree circostanti. Per tale ragione, l'ISPRA ha ritenuto di inviare una nota alle Regioni nella quale, anche in base al principio di precauzione, si sottolinea l'opportunità di assumere provvedimenti cautelativi in occasione della stagione venatoria in corso, fra i quali il divieto di caccia in preapertura, atti ad evitare che popolazioni, ricadenti nei territori interessati da incendi e condizioni climatiche estreme, possano subire ulteriori danni. Con riferimento al rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente ha deciso di affrontare in maniera strutturale le relative problematiche, avviando, in coordinamento con la struttura di missione contro il dissesto, il piano operativo nazionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per il periodo 2014-2020. Tale piano, che è volto alla è volto alla identificazione di un parco progetti, raccoglie il fabbisogno manifestato dalle Regioni, attraverso il sistema Rendis-web. La piattaforma è gestita da ISPRA e, ad oggi, contiene 8.852 proposte di intervento per un totale di 29.520 miliardi di euro. Ad ogni modo, si precisa che l'inserimento di un intervento nella citata banca dati non rappresenta, di per sé, garanzia di finanziamento, ma una condizione necessaria affinché l'intervento proposto possa essere valutato, secondo le modalità ed i criteri fissati dal decreto del ai fini di un eventuale inserimento in future programmazioni, subordinatamente all'accertamento dell'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto ed al superamento della concorrenza con altre richieste segnalate per analoghe finalità. Sempre in tema di dissesto idrogeologico, si segnala che l'ISPRA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati in materia di difesa del suolo, realizza, in collaborazione con le Regioni e Province autonome, l'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI) che contiene ad oggi oltre 614.000 frane, verificatesi sul territorio nazionale. L'ISPRA realizza, altresì, le mosaicature nazionali della pericolosità da frana - piani di assetto idrogeologico (PAI) e gli indicatori nazionali di rischio idrogeologico che forniscono un quadro ufficiale di riferimento sul rischio per frane e alluvioni in Italia e un importante strumento a supporto delle politiche di mitigazione. Si fa presente, da ultimo, con riferimento all'ipotesi di istituzione di una Direzione generale forestale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, secondo quanto riferito dall'amministrazione medesima,

Presidente, intanto non mi ritengo del tutto soddisfatta di questa risposta, sebbene per alcuni aspetti si intravveda,

ha dovuto fare un passo indietro e concludere un accordo per restituire al Corpo forestale il compito di intervenire nel coordinare i Vigili del fuoco, come si era sempre fatto in precedenza.

alimentari e forestali per aggiornare il censimento degli alberi e degli uliveti monumentali e attuare politiche nazionali collegate agli incendi boschivi, è stata istituita solo il 2 ottobre.

l'atto di sindacato ispettivo presentato dalla senatrice Ginetti ci consente di fare un quadro su tutta una serie di riforme

Nell'interrogazione in oggetto si parla di interventi di giurisdizionalizzazione delle controversie, di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte degli uffici giudiziari e di tutto il progetto di informatizzazione della giustizia.

di illustrare compiutamente gli esiti della complessiva azione di ammodernamento avviata negli ultimi anni dal Ministero della giustizia, nella piena consapevolezza che la crescita del nostro Paese passi necessariamente anche attraverso un sistema giudiziario efficiente e rapido nella risposta agli utenti. In tale prospettiva l'informatizzazione e l'uso delle moderne tecnologie nella giurisdizione hanno rivestito un ruolo prioritario nelle politiche del Governo e del Ministero della giustizia in particolare. A distanza di tre anni dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà del processo civile telematico per le cause iscritte avanti ai tribunali di tutta Italia, i risultati conseguiti sono tali da far ritenere ormai acquisito il dato culturale dell'assoluta imprescindibilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per assicurare una giustizia connotata da elevati livelli qualitativi supportata da un'amministrazione in grado di fornire servizi innovativi all'intera cittadinanza, oltre che alle parti dei singoli procedimenti. Il bilancio di tre anni di obbligatorietà fornisce infatti un quadro positivo dell'uso quotidiano della piattaforma. Vorrei fornire alla signoria vostra alcuni dati: dal primo luglio 2014 al 30 giugno 2017 sono stati depositati, da parte di avvocati e altri professionisti abilitati, quasi 20 milioni di atti, in costante crescita di anno in anno. È, inoltre, confermata, la convinta adesione della magistratura all'uso attivo della piattaforma, come testimoniato

hanno raggiunto e superato i 50 milioni, consentendo, negli ultimi tre anni, un risparmio stimato in 178 milioni di euro. L'Amministrazione della giustizia è stata inoltre pioniera nella definizione e nella prima sperimentazione del sistema di pagamento telematico denominato PagoPA. Il successo del servizio è testimoniato dal numero di pagamenti eseguiti sul portale dei servizi telematici, circa 340.000 dal luglio 2014, con un incasso totale prossimo ai 70 milioni di euro. Proprio nella direzione auspicata dalla senatrice Ginetti, giova rilevare che l'insieme dei servizi offerti dalla piattaforma del processo telematico ha portato ad una tangibile riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti monitori, caratterizzati dalla piena telematizzazione, in regime di obbligatorietà anche per quanto riguarda i provvedimenti dei magistrati. In questo campo si è registrata - soprattutto presso i tribunali di maggiori dimensioni - una riduzione della media dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi, rispetto al periodo antecedente l'entrata in vigore del processo civile telematico, oscillante tra il 22

in una fonte di informazioni utili per gli investitori, con particolare riguardo a quelli interessati al settore dei crediti deteriorati L'anno in corso ha infatti visto la definitiva messa in opera, a partire dal mese di luglio, del portale delle vendite pubbliche, un *marketplace* unico nazionale per la pubblicazione e la messa in vendita di tutti i beni, mobili e immobili, di tutte le procedure, un luogo virtuale in cui i beni sono resi più

Sono in fase di ultimazione le attività necessarie alla messa in opera del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi (cosiddetto portale dei creditori, di cui al decreto-legge che ha avuto ad oggetto l'intervento sulle banche). Sono così state poste le basi del sistema Common (*competition money*), attraverso il quale si mira a fornire un ulteriore strumento di valorizzazione dei crediti deteriorati, in modo da trasformare la giustizia civile in volano per l'economia. Il processo di integrale digitalizzazione di tutti i procedimenti civili è ancora in corso con l'obiettivo di estendere la piattaforma del processo civile telematico anche agli uffici del giudice di pace. Merita inoltre segnalare che le politiche di informatizzazione, sulla scorta della positiva esperienza maturata nel settore civile, hanno interessato anche la giustizia penale. È stata infatti completata la diffusione del sistema informativo della cognizione penale (SICP) presso tutti gli uffici giudiziari di primo e secondo grado, a cui ha fatto seguito un'opera di consolidamento dei sistemi, di evoluzione e integrazione degli applicativi. In particolare, è stata avviata la diffusione della funzionalità atti e documenti (A&D) del sistema ed è iniziato il dispiegamento del sistema informativo dell'esecuzione penale (SIES), al fine di conseguire l'automazione di tutte le attività connesse all'esecuzione di una pena inflitta con sentenza divenuta irrevocabile e, pertanto, esecutiva. Dallo scorso mese di luglio è pienamente funzionale l'albo telematico degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati. È ormai in fase di collaudo, e, quindi, sarà messo a breve in esercizio l'applicativo P@ss, per il rilascio in via telematica dei certificati attestanti le iscrizioni, nei registri in dotazione agli uffici di procura, dei procedimenti in fase di indagini preliminari. In questo modo, sarà possibile per il difensore richiedere il certificato di proprio interesse e scaricarlo senza necessità di recarsi presso l'ufficio competente. Sempre nell'ottica dell'efficientamento del sistema giudiziario e del conseguente risparmio di spesa, si collocano le misure assunte per l'implementazione del sistema delle tecnologie necessarie a garantire la partecipazione a distanza nei processi (videoconferenza) e che nell'anno 2018, anche in attuazione delle modifiche normative introdotte con la legge di riforma penale, dovranno essere ulteriormente potenziate. Il complesso delle misure di consolidamento e progressiva evoluzione dei sistemi pone le basi per la realizzazione del processo penale telematico, che tenga conto della particolare delicatezza delle posizioni soggettive coinvolte, oltre che degli aspetti connessi alla sicurezza dei dati e al loro trattamento. In proposito, merita rilevare che la competente direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ha in corso un piano di rafforzamento infrastrutturale delle attività connesse con le intercettazioni che vede la sua prima attuazione nell'acquisto di *server* dedicati e che dovrà essere pienamente dispiegato. In tale contesto, l'alto grado di consapevolezza raggiunto in merito alla sicurezza informatica ha portato a imprimere una decisa accelerazione ai lavori per la realizzazione di una rete protetta per le operazioni d'intercettazione che potrà trovare concreta realizzazione anche grazie all'utilizzo di risorse tratte dal fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio per l'anno 2017. In ordine poi a quanto rilevato dalla senatrice interrogante circa l'opportunità di implementare una banca dati nazionale

ha ultimato tutte le attività per la realizzazione di tale progetto e si è ora in fase di dispiegamento dell'infrastruttura sul territorio nazionale. Sul punto, tra l'altro, lo stesso CSM, con la 7a Commissione, ha adottato tutta una serie di criteri e ha creato un gruppo di studio che sta lavorando proprio sulla banca dati della giurisprudenza di merito. Sono temi che comunque anche nel comitato paritetico Ministero-CSM sono affrontati e seguiti con grande attenzione, efficienza e sinergia. Più in generale, va evidenziato che le politiche d'informatizzazione hanno riguardato la stessa organizzazione del Ministero della giustizia. Nel corso degli ultimi anni, è stata infatti intrapresa un'opera di complessiva reingegnerizzazione dei sistemi informatici del Ministero, accompagnata dalla ricerca di moduli organizzativi idonei ed efficaci a una gestione digitalizzata dei flussi documentali delle varie articolazioni ministeriali, anche al fine di dare piena attuazione al codice dell'amministrazione digitale. In coerenza con tale nuovo e moderno assetto organizzativo, si sta intervenendo anche sulla formazione del personale amministrativo in servizio presso le sedi ministeriali e gli uffici giudiziari, garantendo cicli di addestramento in materia di uso degli applicativi. Il Ministero inoltre, attraverso le proprie strutture tecniche periferiche (coordinamenti interdistrettuali sistemi informativi automatizzati) monitora periodicamente l'utilizzo degli strumenti informatici da parte degli uffici e cura l'assistenza, la formazione dei giudici e dei cancellieri, nonché l'adeguatezza degli strumenti tecnologici. Con riguardo al processo d'informatizzazione della giustizia amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei ministri, interpellata al riguardo, evidenzia come, nel corso degli ultimi quattro anni, il sito istituzionale della giustizia amministrativa sia completamente mutato e, in particolare, oggi non solo è possibile ritrovare

inoltre che il sito istituzionale è arricchito da due speciali, uno dedicato alla cosiddetta riforma Madia, l'altro al nuovo codice dei contratti pubblici. Nel sito ufficiale sono poi pubblicati anche studi dottrinari di massimi studiosi del diritto amministrativo. La rilevanza istituzionale che ha assunto in questi ultimi tempi il sito istituzionale della giustizia amministrativa trova, peraltro, conferma, come riferito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel continuo aumento degli accessi, che sono quasi raddoppiati rispetto alla stessa data dello scorso anno, fino a superare i 500.000 al mese. Il complesso delle iniziative intraprese e i risultati raggiunti testimoniano la massima attenzione riservata dal Ministero della giustizia al tema della informatizzazione della giustizia e consegnano un quadro dell'attuale sistema giudiziario efficiente e rapido, in linea con gli *standard* europei, volano e non più freno per l'economia e la crescita del nostro Paese, come auspicato nell'interrogazione. Quindi, ben venga perché sicuramente sarà nostro dovere - e ci impegneremo in tal senso - continuare su questa strada e portare risultati sempre più soddisfacenti per i cittadini.

Riteniamo, infatti - mi fa molto piacere verificare che anche il Governo ha lavorato in questa direzione - che il potenziamento dei sistemi di informatizzazione e l'introduzione di sistemi ITC in generale

una credibilità nell'ambito di quelle classifiche che all'inizio del 2013 ci vedevano in posizioni di svantaggio. Oggi, grazie a a quanto il Governo ci ha creduto, alle leggi di stabilità che hanno stanziato risorse, possiamo migliorare la nostra posizione e quindi ritenere e quindi ritenere che il sistema giustizia in effetti costituisce, nell'ambito del Paese ma anche nell'Unione europea, un importante volano di sviluppo economico, perché dove la giustizia funziona, in particolare quella civile, gli investimenti e gli investitori si affacciano più facilmente. più facilmente. Mi fa molto piacere il fatto che il processo di informatizzazione possa riguardare anche il sistema penale e che, anche dal punto di vista della giustizia amministrativa, sia stato fatto molto in questa direzione.